A tale proposito, questo Ministero, anche attraverso l'attenta sorveglianza degli uffici territoriali, segue da anni e con la massima attenzione l'evolversi della situazione. Più volte, in vari incontri e manifestazioni, nonché nelle comunicazioni agli organi di stampa, la locale Sovrintendenza ha lamentato la difficile situazione che riguarda tutti gli aspetti della tutela e della fruizione del complesso monumentale, continuando tuttavia a svolgere un'azione di controllo puntuale sullo stato del monumento, effettuando i sopralluoghi periodici, in accordo con le forze dell'ordine e con gli altri enti territoriali, quali la prefettura di Caserta, e con il coinvolgimento del comando dei carabinieri e del comando tutela patrimonio culturale. Nell'ultimo decennio si sono susseguiti interventi di restauro che hanno riguardato la palazzina reale e le due ali laterali, eseguiti in alcuni casi anche con procedure d'urgenza, volti ad arginare la curva di degrado dell'intero complesso. Un ulteriore intervento più recente è ancora in corso di esecuzione ed è mirato al recupero della torre ottagona occidentale che conserva un'importantissima copertura lignea originale ancora *in situ*. Per quanto concerne la questione connessa alla procedura d'asta, la Soprintendenza competente e la direzione regionale, con il supporto dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, hanno attivato ogni misura atta a garantire che l'alienazione del complesso venga sottoposta all'autorizzazione prevista dall'articolo 56 del codice dei beni culturali e del paesaggio onde assicurare, per quanto possibile, la salvaguardia e la tutela del sito reale. Vorrei segnalare che le procedure previste dagli articoli 60, 61 e 62 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che consentono l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero, della Regione e di altri enti pubblici territoriali, possono essere attivate solo successivamente alla stipula di un atto di compravendita, sempre che sussistano, naturalmente, le condizioni finanziarie. Questo Ministero, pur non ignorando la grave situazione economica in cui versa attualmente il Paese, non può che condividere comunque qualunque proposta che miri a consentire il proseguimento della sua attività istituzionale in merito ai più necessari interventi di recupero di un complesso che rappresenta uno degli esempi più ricchi dell'architettura dell'età borbonica.

ma anche perché sono state poste in essere tutte le procedure di tutela previste per la fase di alienazione del bene. Accogliamo anche con favore la proposta della Sottosegretario relativa ad una condivisione degli interventi previsti per il futuro di quest'opera,

il senatore Bianco ed altri senatori richiamano l'attenzione sulla paventata sospensione, disposta dall'INPS, delle visite fiscali d'ufficio per le assenze per malattia dei lavoratori del settore privato, nonché sulle conseguenze di tale determinazione sull'attività lavorativa dei medici che finora hanno svolto tale funzione di accertamento per conto dell'istituto. su esplicita richiesta del Ministero che rappresento, ha comunicato di non aver mai sospeso tali controlli ma di avere solamente previsto, per l'anno in corso, una temporanea riduzione delle visite mediche disposte d'ufficio. Tale determinazione trova la propria giustificazione nelle recenti disposizioni normative che impongono importanti tagli alle spese di funzionamento degli enti pubblici di assistenza e previdenza. In particolare, l'articolo 1, comma 108, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha imposto all'INPS tagli alle proprie spese di funzionamento tali da conseguire, a decorrere dal 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui. L'INPS ha inoltre precisato che, nel corso del 2012, su un totale poco superiore ad 1.200.000 visite mediche di controllo, circa 917.000 sono state disposte d'ufficio, per una spesa complessiva pari a circa 50 milioni di euro, e che all'esito di tali visite è stato possibile pervenire ad una riduzione della prognosi solo in 83.000 casi. Pertanto, alla luce di tali risultanze, l'INPS si è determinato ad incrementare l'efficienza dei controlli medici attraverso una più attenta selezione dei casi da monitorare, pur in presenza di una sensibile diminuzione del numero di visite mediche eseguite d'ufficio. Tale decisione risulta, peraltro, in linea con l'esigenza di una sempre maggiore efficienza dell'azione amministrativa, cui l'INPS ha potuto fare fronte anche mediante l'utilizzo di innovativi strumenti tecnologici, quali ad esempio un sistema di *data mining*, attraverso il quale la scelta dei soggetti da sottoporre a visita di controllo viene guidata da un sistema informatico esperto, che garantisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate. Infatti, attraverso la costante elaborazione di tutti i certificati acquisiti e storicizzati presenti nei *database* centrali, l'istituto è in grado di individuare tutti quelli in costanza di prognosi. In tal senso, il modello di analisi delle certificazioni di malattia è basato su una particolare tecnica statistica di analisi che permette di segnalare i certificati più a rischio in termini di adeguatezza della prognosi, sulla base di un indicatore di probabilità. ricorso alle cosiddette valigette informatiche, di cui sono dotati i medici di controllo, per la redazione - presso il domicilio del lavoratore - del verbale informatico, che viene trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell'istituto. In tal modo l'esito della visita risulta immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile. Il terzo strumento è una nuova procedura, denominata SAVIO, ancora in fase di rilascio, per l'ottimizzazione dell'assegnazione delle visite ai medici di lista. L'INPS ha altresì reso noto di aver valutato il rischio di un possibile incremento della spesa per l'indennità di malattia, come conseguenza della riduzione delle visite mediche di controllo. Al riguardo, l'istituto ha fatto presente, da un lato, che le assenze per malattia dei lavoratori devono essere sempre giustificate dalla presenza di un certificato medico - che si presume essere veritiero in ordine al riscontro dello stato di malattia e, dall'altro, di aver predisposto sia a livello territoriale che nazionale un attento monitoraggio delle visite mediche, attraverso il quale potranno essere rilevate eventuali anomalie circa l'andamento della spesa per la gestione delle visite mediche in oggetto. Proprio in considerazione di ciò, tengo a ribadire che l'istituto ha previsto che la riduzione delle visite disposte d'ufficio riveste solo carattere temporaneo. Per quanto concerne, invece, la ridefinizione dell'attuale tipologia di rapporto di lavoro intercorrente tra l'INPS e i medici fiscali, secondo una prospettiva di stabilizzazione dei medesimi, l'istituto ha precisato che, con i decreti ministeriali del 15 luglio 1986 e del 18 aprile 1996, emanati in attuazione del decreto-legge n. 463 del 1983, viene confermata «la natura di attività libero-professionale del rapporto di collaborazione fiduciaria che si instaura con l'Istituto e la piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico». Pertanto, una ridefinizione della collaborazione improntata ai canoni di stabilità e certezza non può prescindere da un'analisi dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e, più in generale, dal dettato dell'articolo 97 della Costituzione, che impone la regola del concorso pubblico. Con riferimento alla selezione pubblica in corso per il reclutamento di 998 medici esterni, l'INPS ha confermato che il relativo bando riconosce uno specifico punteggio per l'attività prestata presso la pubblica amministrazione in materia previdenziale ed assistenziale. In conclusione, a conferma dell'attenzione riservata dal Ministero che rappresento per la vicenda in parola, faccio presente che è in corso un confronto con l'INPS volto a cercare soluzioni che possano andare nella direzione di una continuità lavorativa dei medici di cui trattasi e della costituzione di un polo unico delle visite fiscali da gestire con il diretto coinvolgimento delle amministrazioni a vario titolo interessate.

luogo, non siamo di fronte a paventate sospensioni: le visite sono state sospese da due mesi.

1.300 professionisti: sarà pur vero che essi hanno un rapporto libero-professionale, ma mi permetta di avere qualche dubbio su tale interpretazione, perché temo che i rapporti libero‑professionali che durano da vent'anni

può darsi che lo sia, ma, come tutti i sistemi informatici che lavorano dal punto di vista della definizione delle categorie di rischio, esso ha bisogno di essere costantemente informato.

Mi permetto di dire che l'efficacia sulla riduzione delle prognosi dipende anche da come e quando viene segnalata la visita fiscale: se la si segnala e la si fa nell'ultimo giorno di prognosi, è evidente che non si un risultato concreto sul piano della riduzione della prognosi stessa. Mi permetto dunque di sottolineare che siamo in una situazione estremamente difficile:

non hanno potuto professionalizzarsi diversamente e oggi sono in una situazione di gravissima difficoltà. Queste sono le motivazioni in base alle quali

che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria oggetto dell'interrogazione hanno ricevuto i bollettini di pagamento fino all'ultimo trimestre in scadenza che, nel caso delle più recenti posizioni definite, è marzo 2013, con possibilità di pagamento entro la fine del trimestre successivo, ovvero il 30 giugno scorso. Con riferimento al pagamento dei contributi volontari utili al raggiungimento del requisito per la pensione, si ricorda che, in base alla legislazione vigente, la contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre sia versato durante il trimestre successivo. Nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso. Qualora, tuttavia, l'autorizzato intenda coprire un periodo inferiore a quello indicato, sufficiente a raggiungere i requisiti pensionistici a normativa vigente, ovvero i requisiti minimi utili a beneficiare delle normative in materia di salvaguardia del diritto a pensione, potrà, accedendo al portale dei pagamenti del sito dell'istituto, modificare e stampare direttamente i bollettini frazionati e pagare l'importo corrispondente, inferiore a quanto notificato in precedenza. In alternativa, tale operazione potrà essere effettuata anche prendendo contatti con la sede competente o con un patronato di riferimento, per richiedere la predisposizione ed il rilascio di un bollettino di importo adeguato al periodo di copertura desiderato. Con messaggio n. 010406 del 27 giugno scorso le sedi territoriali dell'Istituto sono state interessate a garantire la consueta consulenza a coloro che manifestino la volontà di non pagare l'intero periodo e di limitare il pagamento ai soli contributi necessari per il diritto. Voglio ricordare che i contributi volontari versati sono utili al calcolo della pensione, aumentandone l'importo, e sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il versamento è stato effettuato. Con riferimento alle disposizioni in materia di salvaguardia, si fa presente che è possibile per l'istituto emettere certificazioni di salvaguardia solo in favore dei soggetti i quali si trovino nelle condizioni soggettive e oggettive di cui all'articolo 24 del cosiddetto decreto salva Italia, di cui all'articolo 22 del decreto sulla *spending review* e di cui all'articolo 1, comma 231, della legge di stabilità per il 2013. Resta salva la facoltà da parte del lavoratore cessato a seguito di accordi individuali o collettivi di versare la contribuzione volontaria al fine di essere valutato nel *plafond* della categoria dei lavoratori prosecutori volontari, ferma restando la sussistenza di tutte le condizioni di legge previste per quest'ultima categoria. Voglio evidenziare, infine, che nell'ipotesi che il prosecutore versi contributi volontari relativi a periodi che si collocano temporalmente oltre la decorrenza della pensione, l'istituto ha assicurato che procederà d'ufficio al rimborso della contribuzione.

con molto rammarico, devo dichiararmi insoddisfatta rispetto alla risposta ora ascoltata all'interrogazione presentata

È evidente che il problema è grande, direi gigantesco, prodotto da una riforma che, se ha determinato delle positività,

quella di cui parliamo oggi, i cosiddetti prosecutori volontari, fa comprendere che la popolazione italiana, o almeno questa porzione, è stata suddivisa in decine di categorie che,

non si ritenesse opportuno assicurare questi lavoratori che ancora non fruiscono delle garanzie previste dai pacchetti di salvaguardia. Anche al riguardo la risposta non è stata sufficientemente

nonché a predisporre un nuovo sistema di reclutamento ed un piano straordinario di assunzioni. Ricordo che il tema illustrato dagli interroganti è già stato trattato in una serie di recenti atti di sindacato ispettivo, ai quali è stato fornito riscontro durante il mese scorso. Anche in questa sede, però, giova ricordare che con la legge finanziaria n. 296 del 2006 è stato chiuso il canale di reclutamento costituito dalle graduatorie permanenti, trasformando le stesse in graduatorie ad esaurimento. Il successivo decreto-legge 1° settembre 2008, Il successivo decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, ha previsto l'inserimento nelle graduatorie di coloro che hanno frequentato i cosiddetti corsi SSIS

I suddetti corsi - quelli biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico - così come i corsi biennali per la formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento musicale nella scuola media, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, hanno continuato ad essere attivati anche negli anni successivi. Ciò a differenza delle SSIS che sono state invece sospese.

dove far confluire i diplomati dei suddetti corsi negli anni accademici dal 2008-2009 al 2010-2011, assicurando in tal modo a questi ultimi un adeguato sbocco professionale. non sarebbe stato possibile collocarli da nessuna altra parte. La fissazione dell'anno accademico 2010-2011 come termine ultimo per il conseguimento del titolo

Come anche evidenziato nelle precedenti occasioni, il Ministro, in sede di audizione sulle linee programmatiche davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato, ha annunciato l'avvio di un'attenta riflessione sul sistema dì formazione iniziale e sul reclutamento del personale docente. Quanto al personale precario, nella medesima audizione è stata sottolineata l'intenzione di elaborare un nuovo piano triennale di assunzione in ruolo per il 2014-2017 per assicurare l'assorbimento di parte del personale che presta servizio nella scuola con contratti a tempo determinato.

però, che sono parzialmente soddisfatta, perché il Sottosegretario ci ha dato delle informazioni non proprio puntuali. Noi non mettiamo in discussione le intenzioni della ministra Carrozza, con la quale abbiamo avuto modo in in audizione in Commissione di parlare del nuovo piano, e sappiamo che ha a cuore - ed è uno dei suoi punti programmatici - il tema del precariato e della scuola, ma anche di pensare a una risistemazione di tutto il settore. Ciò perché in questi anni ogni Ministro che si è succeduto ha purtroppo introdotto sistemi formativi per l'abilitazione all'insegnamento sempre diversi, producendo delle modalità plurali di accesso che non sempre si sono trasformate in immissioni in ruolo, ma piuttosto hanno contribuito a creare ulteriori categorie di

quando nel 2011 sono state aggiornate le graduatorie ad esaurimento del personale docente in realtà sono state escluse intere categorie di abilitanti e abilitandi dal 2008 in poi. Questo a meno che lei oggi non ci dia la notizia che invece sono stati inseriti anche quelli del 2008, 2009, 2010 e 2011. Tra l'altro, c'è un'anomalia grandissima, perché, mentre si dichiarava di fare delle graduatorie ad esaurimento proprio per mettere fine

create altre figure di insegnanti con il titolo di specializzazione, ma senza possibilità di accedere all'insegnamento. Ci consideriamo pertanto parzialmente soddisfatti, perché dai dati in nostro possesso gli abilitanti del 2009, 2010 e 2011 ad oggi non sono ammessi in questa categoria. Chiediamo quindi al Ministero di farsi carico di questo problema ancor prima di affrontare una nuova sistemazione di tutto il comparto e di trovare soluzioni attraverso attraverso un sistema di reclutamento o un piano straordinario di assunzioni. Noi crediamo che la grande quantità di insegnanti precari presenti nel mondo dell'istruzione

Signora Presidente, la senatrice Lanzillotta chiede una serie di notizie sull'Istituto statale per sordi di Roma. Domanda in particolare la senatrice quali siano i tempi di definizione del regolamento di riordino, quale sia la posizione giuridica del commissario straordinario e solleva perplessità sulla costruzione di un parcheggio multipiano sotterraneo all'edificio, auspicando che il Ministero intervenga per sospendere l'iniziativa. Quanto alla richiesta sullo stato di elaborazione e sui tempi di approvazione del regolamento di riordino dell'Istituto, occorre prima di tutto ricordare che una prima stesura dello stesso non fu ammessa a registrazione dalla Corte dei conti nel 2004. La procedura fu puoi riattivata dal MIUR nel 2007, con la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze di un nuova versione, che teneva conto di tutte le osservazioni a suo tempo mosse anche dalla Corte dei conti. Il Ministero dell'economia e delle finanze si espresse però ancora una volta sfavorevolmente, non tanto sui contenuti del regolamento, quanto sull'opportunità della sua adozione, ritenendo l'iniziativa in controtendenza con la linea politico‑finanziaria di contenimento della spesa pubblica ormai da tempo perseguita anche allora dal Governo, ispirata ad una drastica riduzione del numero degli enti pubblici. L'iniziativa è stata ripresa nel 2009 con la riproposizione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte del MIUR di un ulteriore schema di regolamento, ma anche in questa occasione il suddetto Dicastero ha ribadito la propria contrarietà. Tutto ciò non sottintende che la volontà del MIUR non sia ancora quella di portare a termine il processo di riordino. riordino. C'è l'impegno da parte di questo Ministero a riprendere il tema, anche con il MEF, per trovare una soluzione e dare attuazione ad una legge dello Stato. Relativamente alla posizione del commissario straordinario, professor Ivano Spano, quest'ultimo è stato designato con decreto del Ministro nel 2007. Nessuna ipotesi di lavoro, senatrice Lanzillotta, è oggi allo studio da parte del Ministero. Ci ragioneremo in tempi brevi e sarà quella l'occasione per verificare anche la posizione del professor Ivano Spano, che, come lei afferma giustamente nella sua interrogazione, è stato designato già nel 2007. Nella seconda parte dell'atto di sindacato ispettivo l'interrogante illustra con dettaglio il piano di costruzione di un parcheggio multipiano seminterrato sul terreno di proprietà dell'Istituto e solleva una serie di perplessità sull'impatto che tale iniziativa potrebbe avere sulle ordinarie attività didattiche, sugli utenti e anche sul contesto urbanistico di riferimento. Il Ministero condivide quanto rappresentato. Non vi sono dubbi che, considerata l'entità dell'intervento in programma (si parla di più livelli sotterranei di parcheggio) e il protrarsi dei lavori edilizi per un lungo periodo di tempo, ne verranno gravemente compromesse le attività dell'Istituto e il benessere psicofisico di tutti gli utenti. È facilmente immaginabile come durante i lavori non potranno essere pienamente utilizzate le strutture destinate alla didattica e alle attività connesse e come l'espletamento delle medesime attività, in un contesto che, a causa degli effetti collaterali dei lavori di scavo del sottosuolo, vede compromessa la salubrità ambientale, risulti oltremodo pericoloso. L'avvio dei lavori precluderà poi agli utenti dell'Istituto l'utilizzo dell'unico spazio verde disponibile, circostanza tanto più grave in quanto ad usufruire di tale spazio sono soprattutto i bambini, molti dei quali - ricordo - a ridotta capacità di interazione con l'ambiente sociale. Per queste ragioni il Ministero assicura tutto il sostegno del caso, con l'eventuale avvio anche di un tavolo tecnico per individuare modalità di finanziamento diverse dell'Istituto, che non incidano in termini così negativi sulle attività didattiche e sulle strutture a ciò predisposte. Medesima rassicurazione è fornita sull'adozione di tutte le iniziative di competenza per scongiurare il verificarsi dei problemi illustrati dall'onorevole interrogante.

la funzionalità di un istituto che è unico nella capitale, e in particolare l'attività di integrazione e inclusione tra bambini non udenti, bambini plurihandicap e bambini udenti,

Signora Presidente, le interrogazioni propongono un tema al centro dell'attenzione del Governo in questo momento. La vicenda della Berco è segnata da una situazione produttiva e occupazionale che è andata via via peggiorando negli ultimi anni. Già con decreto 26 agosto 2010, su richiesta dell'azienda, il Ministero del lavoro approvava un primo piano di ristrutturazione, presentato all'epoca, autorizzando nel contempo la corresponsione, a decorrere dal 1° maggio 2010, del trattamento di cassa integrazione straordinaria per 24 mesi per un massimo di 2.609 unità lavorative in forza presso i tre stabilimenti della Berco: Copparo, in provincia di Ferrara, Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso e Bussano, in provincia di Torino. Successivamente, in considerazione della particolare complessità dei processi produttivi attivati e della permanenza di una eccedenza di personale, il Ministero del lavoro ha concesso, il 30 ottobre 2012, la proroga del programma di ristrutturazione fino al 30 aprile 2013, autorizzando un'ulteriore corresponsione del trattamento di cassa integrazione straordinaria.

A seguito di questa iniziativa dell'azienda, il Ministero dello sviluppo economico, in accordo con il Ministero del lavoro, ha condotto una serie di incontri sia con l'azienda stessa sia con i sindacati, al fine di esaminare le questioni sollevate proprio dagli interroganti e la complessità della crisi. Proprio nei giorni scorsi si è tenuto ancora un incontro nel quale erano presenti i rappresentanti delle istituzioni territoriali

da un lato con le parti sociali e dall'altro con l'azienda, sulle prospettive economiche e occupazionali della Berco, finalizzato alla ricerca di una possibile intesa sulla soluzione della crisi. Da ultimo, il Ministero del lavoro, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato per il prossimo 9 luglio luglio il tavolo con l'azienda e i sindacati per l'esame della procedura di mobilità, ma all'interno di questo è intenzione dei due Ministeri chiedere all'azienda di chiarire fino in fondo il proprio piano industriale, chiarire le prospettive produttive e di posizionamento di mercato della Berco e, in funzione di questo, fare un ragionamento su quali siano gli ammortizzatori sociali più utili per gestire la situazione; non diamo, cioè, per scontato che la procedura di mobilità sia l'unico strumento possibile. Segnalo che la società opera nel settore delle macchine movimento terra agricole (in particolare costruisce i cingoli), e da questo punto di vista è una delle imprese *leader* a livello mondiale, in particolare sul sul cosiddetto mercato libero, cioè là dove si produce per terzi. Per capirci, la principale impresa del settore a livello mondiale è la Caterpillar, ma quest'ultima produce largamente in condizioni di integrazione verticale, quindi fornendo cingoli alle proprie macchine. Invece la Berco, come altre società, produce cingoli per terzi ed è una delle società *leader* a livello mondiale. Quindi, il Governo giudica il futuro della Berco estremamente importante per il nostro Paese, oltre che naturalmente per le aree territoriali in cui sono siti gli stabilimenti. La Berco ha subìto un deterioramento molto pesante delle proprie condizioni economiche e finanziarie e una contrazione dell'attività certamente in conseguenza della crisi economica complessiva che attraversa

anche tenuto conto che la Berco ha perso quote di mercato e quindi ha perso posizioni sul mercato. Questo processo è andato aggravandosi nel corso del 2012 e in questo inizio di 2013. Quindi, la situazione è molto complessa e difficile. Il Governo ritiene la Berco un'azienda di importanza fondamentale per il nostro Paese, per cui il punto chiave è come ridisegnare una strategia industriale dell'azienda che dia un futuro produttivo e competitivo alla Berco; all'interno di questa potranno essere attivati gli ammortizzatori sociali migliori da questo punto di vista. Potrò aggiornare gli onorevoli interroganti dopo l'incontro del 9 luglio, che - ripeto - è molto importante proprio per chiarire le prospettive della Berco.

sia l'importanza dell'azienda che il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali proprio per l'importanza che essa ricopre nell'economia della Provincia di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna hanno consentito a tutti gli attori coinvolti di seguire il processo che oggi lei ha in modo puntuale riportato

il riconoscimento dell'importanza strategica che un'azienda di queste dimensioni ha per l'economia non di Ferrara, non dell'Emilia-Romagna, ma dell'intero Paese,

necessario, riproporrò assieme agli altri firmatari un'altra interrogazione che le consenta di tornare in quest'Aula ad aggiornarci dopo la data, che aspettavamo da tanto tempo, del 9 luglio, giorno in cui finalmente l'azienda dovrà sedersi a quel tavolo a cui a tutt'oggi o non si è presentata o lo ha fatto in modo separato rispetto agli altri attori, preferendo tavoli diversi. diversi. Il tema vero, come lei ha detto, è l'incombenza della procedura di mobilità che è stata aperta nei fatti l'8 maggio, a poche ore da un incontro che, invece, aveva lasciato presagire l'apertura di una trattativa con le parti sociali, che non è avvenuta. È stata quasi la risposta a quell'incontro, ed è una procedura che scade il 22 luglio;

ha nel proprio destino questa azienda. Il nodo vero è che non abbiamo ancora visto nessun piano industriale; non sappiamo se c'è un'intenzione di vendita

interessi e quali tipi di interesse potessero essere stati manifestati nei confronti dell'azienda. Le possibilità di vendita non si sono realizzate e, a tutt'oggi, non sappiamo effettivamente

Vi è stata una prima apertura da parte del direttore generale del personale della Thyssen, a dire: noi confidiamo molto nel ruolo di intermediazione del Governo in questa vicenda e ci facciamo portatori, anche nei confronti dell'amministratore delegato, affinché venga favorita l'apertura della trattativa a titolo che il 22 luglio di fatto venga tolto di mezzo e si consenta l'apertura di una trattativa che

realtà della zona del trevigiano e, in particolare, del Comune di Castelfranco Veneto. Prendo atto, come la collega che mi ha preceduto, della ricostruzione che è stata fatta, la quale dà conto dei passi avanti compiuti nel tentativo di far dialogare i vertici aziendali con le parti sociali e gli organi istituzionali nell'ambito del Ministero, proprio perché la preoccupazione che ad oggi avvertiamo è quella che, purtroppo, lo stato di fatto ci racconta: una situazione di

Pertanto, posso ritenermi parzialmente soddisfatta di questa risposta, perché apprezzo il tentativo che il Ministero ha messo in campo di intavolare discussioni più serie tra parti sociali e - ribadisco - i vertici aziendali, che hanno disertato le ultime occasioni. occasioni. Auspico veramente che il ministro Zanonato, proprio in quanto conoscitore di questa realtà territoriale, possa pensare e provvedere anche a ragionamenti più ampi che diano maggiori garanzie a questi lavoratori di quelle che possono essere le conseguenze immediate nella loro vita

Ricordo che gli operai dipendenti del ramo aziendale con sede nel mio comune si sono resi disponibili ad alternative, come i contratti di solidarietà, ma è stata proprio l'azienda su questo punto a non mostrarsi molto disponibile all'ascolto. Credo, tuttavia, che il Governo debba fare molto di più. Mi fa piacere che lei abbia sottolineato che il Ministero abbia conoscenza e coscienza del ruolo importante e strategico che l'azienda ricopre, non solo per l'area veneta e per la zona territoriale del trevigiano e del Comune di Castelfranco, ma per l'intero Paese. Vorrei ricordare che è un'area produttiva che risente di altre situazioni di forte crisi, che tanto dà in termini di contributo non solo lavorativo, ma anche economico, produttivo e sociale al resto del Paese, ma che, come contropartita, purtroppo ottiene poco. Auspico che nell'incontro del 9 luglio si possa affrontare un ragionamento di più lungo respiro che dia conto anche dell'intenzione del Governo di adottare politiche economiche e industriali diverse. In questo momento, nel nostro Paese sono assenti e io assisto ad una sorta di immobilismo sotto questo profilo.

Il Governo sta seguendo con grande attenzione il processo di riorganizzazione e di rilancio delle attività delle aziende del gruppo. Il nuovo gruppo dirigente di Finmeccanica ha affrontato e sta affrontando complesse situazioni di mercato che richiedono iniziative rapide per migliorare la competitività e superare gli squilibri che ancora permangono.

Il programma valorizza i settori e le aziende nei quali Finmeccanica eccelle, a cominciare da aeronautica, elicotteristica, elettronica applicata alle tecnologie satellitari e alle telecomunicazioni, sistemi di controllo delle reti di trasporto e di energia, apparati per la produzione di energia elettrica elettrica tradizionali e nucleari, eccetera. La focalizzazione che è in corso non significa che il settore civile non abbia un futuro importante all'interno di Finmeccanica. Noi crediamo che ci siano spazi per un futuro del settore civile. È certo però che c'è bisogno di chiarire meglio il *core business* di Finmeccanica e anche di dare nel settore civile - ma in particolare sto pensando ad Ansaldo Energia e Ansaldo Breda, due realtà molto importanti di tale settore di Finmeccanica *partnership* anche internazionali che consentano un miglioramento della posizione di mercato di queste due aziende e un loro inserimento all'interno di sinergie internazionali che ne potenzino la competitività e ne allarghino gli sbocchi di mercato.

tecnologie dell'elettronica per la difesa ma anche per sistemi di sicurezza, ed anche per il settore civile. Selex ES, cioè Selex electronic systems, nasce il 1° gennaio di quest'anno attraverso la concentrazione delle attività di Selex Galileo, Selex Elsag e Selex sistemi integrati. L'obiettivo della costituzione di Selex ES è il perseguimento di un migliore posizionamento competitivo nel settore di riferimento e di una concentrazione sui prodotti di maggiore qualità e capacità di penetrazione sul mercato. La dichiarata *vision* della nuova azienda è di essere così un forte punto di riferimento per i clienti e i *partner*, offrendo eccellenza tecnologica nei sistemi elettronici e soluzioni per costituire una «comunità» più sicura e intelligente. Per raggiungere questo obiettivo, Selex ES ha avviato un percorso finalizzato a una politica di investimenti mirata allo sviluppo di nuovi prodotti e al mantenimento di quelli *core*; alla realizzazione di economie di scala necessarie a raggiungere la «massa critica» per competere sul mercato globale; un piano di riorganizzazione aziendale orientato a creare un'azienda snella, efficiente e maggiormente competitiva. Al fine di concretizzare gli orientamenti strategici che ho appena segnalato, l'azienda sta già intervenendo sulle seguenti aree: razionalizzazione del portafoglio prodotti per aumentare la profittabilità, la competitività e la crescita sostenibile della società; ottimizzazione dell'ingegneria e della produzione, focalizzandole su centri di eccellenza ed internalizzando le attività pregiate; efficientamento della politica di acquisti; ottimizzazione delle strutture di *staff*, attualmente distribuite in 39 siti in Italia; razionalizzazione dei siti per evitare la dispersione e le sovrapposizioni esistenti; dimensionamento degli organici, in Italia, con un intervento in due direzioni. L'accorpamento e lo sfruttamento delle economie di scala, economie di scala, con la razionalizzazione dei siti e l'ottimizzazione delle strutture di *staff*, implica una riduzione di risorse lavorative per 840 unità dirette e 1.098 unità indirette nel nostro Paese. Poi ci sono riduzioni anche in altri Paesi, in particolare in Gran Bretagna, che però in questo momento tengo fuori dal quadro che sto descrivendo. In particolare, il piano di ridimensionamento degli organici è condizionato dal raggiungimento dei *target* di acquisizione degli ordini nel periodo di piano 2013-2017. Sulla base del piano industriale e di riorganizzazione di Selex e di questo piano di ridimensionamento degli organici, è cominciato un confronto approfondito con le organizzazioni sindacali. Si è partiti con un accordo di protocollo molto importante, firmato il 20 febbraio scorso, in cui l'azienda si è impegnata a non intraprendere nessuna azione unilaterale senza il preventivo confronto con i sindacati. Si è poi avuto un accordo con Federmanager e la rappresentanza sindacale aziendale dei dirigenti, per la riduzione di 120 dirigenti in tre anni, un accordo per la collocazione in mobilità di 810 unità e uno per la chiusura di quattro siti in Italia. Il confronto sta proseguendo e nelle ultime giornate di giugno è stato firmato un accordo tra azienda e sindacati. Il piano su cui è stata trovata l'intesa prevede 1.610 eccedenze strutturali, che saranno gestite con la mobilità volontaria finalizzata all'accompagnamento alla pensione, con contratti di solidarietà, con la stabilizzazione dei precari. È prevista inoltre, nell'arco di vigenza del piano di riorganizzazione, l'assunzione di 300 giovani con contratti di apprendistato. In altri termini, la gestione delle eccedenze su cui l'azienda si è impegnata avviene mediante l'utilizzazione non solo di ammortizzatori sociali, ma anche di risorse dell'azienda stessa, ad integrazione degli ammortizzatori sociali, in modo da ridurre al minimo l'impatto sulle tutele per i lavoratori coinvolti, quindi per esempio con un forte accento sull'accompagnamento - anche a carico dell'azienda - fino alla pensione, sui contratti di solidarietà e sulla stabilizzazione dei precari. Significativo giudichiamo il fatto che sia previsto un processo di assunzione di 300 giovani con contratti di apprendistato. Nell'annunciare l'accordo, i sindacati hanno espresso un giudizio positivo sul testo complessivo dell'intesa, pur consapevoli dei sacrifici che interessano una parte considerevole dei lavoratori di Selex ES, convinti però che tali sacrifici devono essere finalizzati al risanamento e al rilancio della Selex ES. A noi pare che il piano presentato dall'azienda vada esattamente in questa direzione, quindi con un potenziamento delle capacità competitive della Selex, e dà quindi un contributo molto importante al futuro produttivo dell'azienda.

importante, sia da parte delle organizzazioni sindacali che lo hanno firmato e dei lavoratori che lo devono sostenere, sia, certamente, da parte dell'azienda. Credo che non sfugga a nessuno il fatto che quella tipologia di intesa contiene una scelta

rapidi e stretti, un sostegno vero alla riorganizzazione e agli investimenti di prospettiva strategica.